esteri*. Signor Presidente, l'interrogazione del senatore Selva ci dà l'opportunità di sottolineare che l'Italia segue con grande

In questa riunione sono state affrontate questioni particolarmente sensibili come il rispetto delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla libertà di espressione e di culto, le detenzioni arbitrarie, la tortura, i diritti delle minoranze, la pena di morte, l'abolizione della pena di morte, la ratifica del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966 e la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale. Queste consultazioni forniscono anche l'occasione all'Unione Europea per segnalare alle autorità cinesi casi individuali di detenuti per reati di opinione, di vittime di trattamenti inumani e degradanti e di condannati a morte. L'Unione Europea proprio recentemente ha espresso la propria preoccupazione per gli episodi di intimidazione e repressione nei confronti di cattolici e protestanti. Fra i casi individuali sollevati sistematicamente dalla UE vi sono proprio le vicende a cui lei fa riferimento dei due religiosi, Jia Zhiguo (vescovo cattolico) e Zhang Rongliang (pastore protestante). L'Unione Europea non cessa di cogliere l'occasione di ogni dialogo Europea e Cina per chiedere informazioni a loro riguardo, sollecitandone la liberazione. Alle nostre richieste le autorità cinesi hanno finora risposto negando che, in questi casi, ci si trovi di fronte a fenomeni di persecuzione religiosa. Nel caso di Zhang Rongliang, hanno dichiarato che il pastore protestante era sotto inchiesta con l'accusa di falsificazione di documenti. Nel caso di Jia Zhiguo, le autorità cinesi hanno sostenuto di non aver adottato alcuna misura restrittiva nei suoi confronti. Come già è accaduto negli anni scorsi, né l'Italia né gli altri *partner* comunitari hanno ritenuto queste spiegazioni del tutto soddisfacenti. Si sono riservati pertanto di continuare ad adoperarsi a favore dei due religiosi tanto con passi specifici

Sottolineo inoltre che lo stesso Presidente del Consiglio, nel suo recente incontro in Cina con il Presidente cinese e con il Primo Ministro, ha tenuto a ribadire le posizioni

che abbiamo suggerito alle autorità cinesi, come gesto significativo, di adottare la moratoria sulla pena di morte almeno durante le prossime Olimpiadi del 2008 che si terranno in Cina.

Il Sottosegretario, dalle carte che gli sono state preparate, ha dato una generica indicazione circa i passi che possono essere stati fatti per il rispetto, altrettanto generico, dei diritti umani. Cerco di fornire altri elementi al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, perché quello del vescovo che ho ricordato è solo un caso,

dal Governo, ed una Chiesa in gran parte clandestina, i cui vescovi sono nominati secondo le leggi canoniche e anche civili dal Vaticano.

Altri dieci sono i cosiddetti vescovi sotterranei, quelli che sono stati perseguitati con asprezza in passato. Questa asprezza oggi non è per nulla diminuita.

perché agli arresti, alle uccisioni si accompagna anche un rigoroso mercato di organi prelevati da detenuti cinesi, altra cosa che fa inorridire la nostra coscienza. In Cina avviene il più alto numero di esecuzioni sommarie che in qualunque altro Paese del mondo. Ecco la ragione per cui, signor Presidente, onorevoli membri del Governo (soprattutto, un Governo come questo, che si avvale del sostegno anche di coloro che in altri tempi hanno esaltato il maoismo e ancora portano nel loro emblema e nel loro nome l'espressione "comunista"), credo vi sia una riflessione supplementare da fare quando siamo in presenza di condizioni quali queste in cui si trovano sacerdoti e laici. Per quanto riguarda l'osservazione fatta a proposito di di ciò che il Governo pensa di suggerire in occasione delle Olimpiadi, io avrei tentato la strada che prospetto nella mia interrogazione, ma vedo che, anche se fu tentata ai tempi dell'Argentina,

vengano liberate e, in modo particolare, si accompagni all'azione di tanti altri Paesi la nostra azione determinante per l'eliminazione della pena di morte praticata, come si evince dalle cifre che ho citato, nel modo più ampio e talvolta

Signor Presidente, signor Sottosegretario, le ragioni che mi hanno indotto a presentare il 28 giugno di quest'anno l'interpellanza in esame, che poi mi hanno costretto anche a sollecitarla per ben tre volte,

9 aziende territoriali, di cui una per ciascuna provincia, 17 aziende ospedaliere autonome, 4 di riferimento per l'emergenza di terzo livello e 13 di riferimento per l'emergenza di secondo livello, 3 policlinici universitari, un istituto di carattere scientifico, un ospedale classificato, un istituto presidio di ASL nonché 61 case di cura private accreditate.

e all'inizio di quest'anno, con una serie di fatti che hanno determinato anche l'intervento di interesse non solo del Governo ma anche della magistratura, che hanno portato la Commissione d'inchiesta la Commissione d'inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nella passata legislatura ad esprimere un giudizio molto severo sul funzionamento del servizio sanitario siciliano.

tra le forze politiche del Governo regionale della passata legislatura, che poi è analogo a quello dell'attuale legislatura. Ricordo che la stampa e poi anche la magistratura si occuparono delle nomine operate nel marzo del 2005 allorquando perfino componenti della maggioranza che sosteneva il Governo regionale denunciarono pubblicamente una vergognosa «lottizzazione», una vergognosa «lottizzazione», che non solo caratterizzò la nomina dei direttori generali ma perfino quella dei direttori amministrativi e sanitari. Voglio ricordarle, onorevole Sottosegretario, che le aziende rimasero per mesi senza direttori amministrativi e senza direttori sanitari: questo perché ai direttori generali già nominati non era consentito esercitare la funzione

Detta situazione, tra l'altro, si aggiunge al fatto che la Regione siciliana è quella che ha il più alto numero di case di cura accreditate private (61), che ha 4.642 posti letto di sanità privata accreditata, il cui *deficit* nel settore della sanità nell'anno precedente è stato di circa 650 milioni di euro e che si calcola dovrebbe

2.400 miliardi delle vecchie lire. Quindi, un disavanzo spaventoso per tenere in piedi una struttura

gli specialisti convenzionati della Regione siciliana (non solo di branche a visita ma anche di diagnostica strumentale), un numero da solo superiore, credo, a tutto il resto delle Regioni italiane. Vi è quindi uno strettissimo rapporto tra consenso, potere politico clientelare e sanitario in Sicilia. Ma non vi è solo questo: vi è anche un intreccio tra il sistema sanitario regionale e l'organizzazione criminale mafiosa. Non sono pochi i direttori generali che sono stati coinvolti in indagini della magistratura, alcune anche con riferimento a reati di mafia (tra l'altro, lo stesso Presidente della Regione); non sono pochi i titolari di case di cura private e gli operatori sanitari anche pubblici che sono stati coinvolti in indagini che riguardano il reato di associazione

quella della Provincia in cui abito, che a giudizio della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale fu considerata l'unica Provincia in cui il servizio sanitario funzionava, quindi nell'unico luogo per cui, in qualche maniera, vi era un giudizio positivo, siamo rimasti

effettivamente le funzioni e preso possesso dei propri uffici perché non è stato ancora completato l'*iter* relativo alla loro nomina. Quindi, ancora adesso, quattro aziende sono commissariate con commissari che hanno poteri solo per assolvere agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione in una realtà, come quella siciliana, che ha ha le caratteristiche che mi sono permesso di descrivere. Il senso della mia interpellanza è ovviamente non solo quello di di denunciare questi fatti, ma anche di comprendere le ragioni che hanno impedito al Governo nazionale di esercitare le funzioni che la legge gli attribuisce, cioè di attivare, decorsi i termini perentori - dice la normativa

posto. Se dovesse poi avvenire quanto è avvenuto nel marzo 2005, passeranno mesi affinché questi direttori generali possano nominare i direttori amministrativi e sanitari e quindi si entrerà in una situazione di grande precarietà; il tutto - ripeto - mentre la Regione siciliana sarà chiamata a svolgere una funzione importantissima per allinearsi, sotto il profilo della spesa, alle nuove disposizioni contenute nella finanziaria e a recuperare il *deficit* che la caratterizza. Tra i direttori generali già nominati a marzo nelle altre aziende, ve ne sono ve ne sono alcuni sottoposti a procedimento penale; altri non hanno chiuso il bilancio in pareggio, anzi hanno bilanci assolutamente in notevole e significativo disavanzo;

riferisco ad Aiello - oggi accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono regolarmente in servizio; ve ne sono alcuni nominati e poi dichiarati decaduti perché avevano attestato falsamente il possesso dei requisiti.

Il fatto che vi siano direttori generali che non hanno i requisiti previsti dalla legge è stato ampiamente denunciato dalla prima Commissione legislativa presso l'Assemblea regionale siciliana che ha il compito di

di esperienza di conduzione di strutture complesse. Addirittura per uno di questi è stato talmente evidente che da un anno e mezzo è stato dichiarato decaduto; il che ha portato la prima Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, nel dare il parere sulla nomina di questi direttori generali delle quattro aziende, oggetto dell'interpellanza, a subordinare l'effettiva nomina, l'effettiva stipula del contratto all'accertamento dei requisiti ed a verificare se i nominati abbiano o no procedimenti penali in corso. Tutti sanno che avere procedimenti penali in corso non implica di per sé il fatto di non essere nominabili. Però, in un contesto come quello siciliano, mi chiedo se non sia opportuno evitare che le nomine riguardino soggetti che hanno gravi procedimenti penale in corso. Non solo, ma tra i non confermati nella precedente nomina vi sono i direttori generali, che non sono stati confermati solo perché avevano superato i 65 anni di età. Tra la nomina degli attuali direttori generali sono nominati soggetti che hanno superato i 65 anni di età, dimostrando che il criterio dei 65 anni di età è un criterio che si utilizza a secondo dell'effetto che si vuole determinare. Insomma, Sottosegretario,

alcuni dei quali sono di nomina governativa nazionale e non stanno svolgendo la funzione cui sono chiamati, se è vero, com'è vero, che moltissime aziende hanno chiuso i bilanci in forte disavanzo, non consentita dall'attuale normativa e dall'accordo a suo tempo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Questo era il senso della mia interpellanza. Concludo con il solo rammarico di poterne discutere in Aula oltre tre mesi dalla sua presentazione, nonostante avessi, con diversi solleciti, richiamato l'urgenza di una trattazione in tempi che fossero più consoni alla gravità di quanto oggetto dell'interpellanza stessa.

se lei, con il suo dire circostanziato e molto preciso, vuole coinvolgere me e il Governo in un giudizio talora problematico, spesso poco lusinghiero, sull'organizzazione e la gestione della sanità siciliana, ebbene, preciso con molta sincerità che sfonda una porta aperta. la professione di medico nella sanità pubblica; mi sono sempre occupato di sanità pubblica e conosco perfettamente la situazione della sanità siciliana. Per quanto riguarda il richiamo doveroso e giusto che lei ha fatto alla necessaria vigilanza, che è compito del Ministero e del Governo centrale, in ordine alla tutela della salute in quelle zone e quindi a favore dei

che prevede non una riedizione dei patti precedenti tra Governo e Regioni, ma contiene una forte novità in ordine all'affiancamento e potere del Governo nei confronti delle Regioni che hanno difficoltà strutturali nella spesa e nel rientro dei bilanci. Non c'è solo la Regione siciliana che è in queste condizioni. Altre Regioni molto importanti versano nello stesso stato di grave disagio economico, che poi esprime una difficile, spesso problematica - uso un eufemismo - capacità di governo degli eventi in campo sanitario. Sono convinto che stiamo per dare vita a un corpo tecnicamente valido che avrà anche una cabina di regìa politica allo scopo di affiancare queste Regioni in difficoltà, cui lo Stato dovrebbe garantire

Per fare questo però, ripeto, ci sarà un affiancamento che interverrà sui modi in cui la gestione della sanità in queste Regioni viene esercitata. Spero che questo nuovo strumento ci consenta un intervento molto più attivo di quanto non sia stato

questo atto ispettivo, altrimenti mi sarei premurato in maniera diversa: evidentemente i nostri uffici ci hanno messo con ritardo in condizione di rispondere. ha molti elementi di contenuto giuridico e burocratico e forse non la soddisferà, ma purtroppo corrisponde allo stato dei fatti. La situazione riportata nell'atto parlamentare riguarda l'esercizio dei poteri sostitutivi, previsti dall'art 2, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel caso in cui nelle aziende sanitarie locali o in quelle ospedaliere perduri la gestione di un commissario straordinario di nomina regionale. Poiché l'esercizio dei poteri sostitutivi configura certamente una limitazione dell'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione, è indispensabile la presenza di tutti i presupposti, sia in termini sostanziali che formali, richiesti dalla normativa. L'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto citato richiama la necessità della nomina dei Direttori generali entro il termine perentorio «di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio». Nel caso in esame tale norma va armonizzata con l'articolo 11, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 30 del 3 novembre 1993, il quale stabilisce che «in caso di mancanza del legale rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nelle more della nomina da parte del Presidente della Regione del nuovo titolare, l'assessore regionale per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera». Poiché nei casi segnalati da lei, senatore Battaglia, non rileva la *vacatio*, per la presenza di un commissario di nomina regionale, non si può configurare la possibilità dell'esercizio del potere sostitutivo; inoltre, un'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 2-*octies*, condurrebbe alla nomina di un commissario *ad* *acta*, con analoghi poteri di quello di nomina regionale. Non cambieremmo molto la situazione. Appare, peraltro, auspicabile che in tutti gli enti di gestione della sanità pubblica possa essere garantita la maggiore certezza possibile circa la titolarità degli organi di vertice, allo scopo di assicurare una efficace individuazione e realizzazione delle strategie aziendali. La situazione nella Regione Sicilia - trovo scritto - si è «normalizzata» (posso aggiungere che sembrava si fosse normalizzata) poiché la Giunta regionale di governo e questo è sorprendente - nella seduta del 21 luglio 2006, ha nominato i direttori generali delle Aziende gestite fino a tale data dai commissari straordinari. Sono di seguito elencati i nomi dei nuovi direttori generali. Apprendo adesso, per la prima volta, che questi direttori nominati

Signor Presidente, è del tutto evidente che nell'aver richiamato l'attenzione del Governo sul ritardo con cui l'interpellanza viene riscontrata non vi era ovviamente alcuna critica né al Sottosegretario, che oggi cortesemente, invece, risponde all'interrogazione, né al fatto che questo fosse un avvenimento di particolare rilievo critico. Voglio solo ricordare che, quando si avanza un'interpellanza, normalmente ci si riferisce ad un fatto che sta accadendo in quel momento; se le risposte arrivano dopo tanti mesi il fatto in sé si può già ritenere, talvolta, superato dalle circostanze. D'altronde, se l'interpellanza è svolta da un senatore di maggioranza, che sostiene convintamente il Governo, evidentemente qualcosa da dire

ho contribuito a scrivere, in quanto allora ero Presidente della Commissione sanità dell'Assemblea regionale siciliana, faceva riferimento ad una condizione transitoria e non ad una situazione che poteva protrarsi nel tempo. La stessa nomina dei commissari era a tempo. Nulla impediva al Governo regionale di poter procedere ancor prima della scadenza ad attivare le procedure per la nomina dei nuovi direttori generali. Evidenzio solo che nella risposta non si fa alcun riferimento - non potrebbe essere diversamente essendo una risposta di natura istituzionale - alle circostanze che hanno impedito

una spaventosa lottizzazione, che purtroppo sta proseguendo. Per il resto mi dichiaro soddisfatto e ringrazio il Governo per la risposta.

la pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Lucca risulta allo stato composta da un presidente, due presidenti di sezione e 25 magistrati, per un totale di 28 unità. L'organico, peraltro, presenta la vacanza delle figure del presidente del tribunale, vacanza pubblicata sin dall'11 aprile 2005, e di uno dei presidenti di sezione, vacanza non pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, nonché di tre dei complessivi 23 giudici ordinari, due di queste vacanze pubblicate il 27 dicembre 2005, e infine di uno dei due giudici del lavoro. Anche questa vacanza è stata pubblicata. Le esigenze operative del tribunale di Lucca sono state già oggetto di valutazione in occasione dei primi due interventi di riparazione delle 546 unità di magistrato, recate in aumento dalla legge n. 48 del 2001, disponendosi l'ampliamento della pianta organica in ragione di due posti di giudice. Non si ravvisa pertanto allo stato una situazione di scopertura dell'organico. Per quanto concerne la richiesta di istituzione nella città di Lucca di una sede di corte d'appello o di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, si fa presente che provvedimenti del genere non hanno, come è noto, natura di atto amministrativo ma di atto avente forza di legge, e allo stato non vi sono iniziative in tal senso. Per quanto riguarda invece la diminuzione dei fondi, la situazione del tribunale di Lucca non è per nulla dissimile dalla situazione comune a tutti gli uffici giudiziari, essendo noto che le spese di funzionamento dell'apparato giudiziario hanno subito un'incisiva decurtazione negli ultimi cinque anni, pari al 52 Per quanto riguarda l'assistenza e l'acquisto di materiale per il funzionamento delle fotocopiatrici di proprietà dell'amministrazione, i relativi fondi sono tratti sul capitolo 1468 e vengono assegnati direttamente ai funzionari delegati competenti per territorio che decidono discrezionalmente. Agli uffici giudiziari di Firenze sono stati assegnati i seguenti importi: corte d'appello di Firenze, con tre ordini di accreditamento, 68.600 euro, a fronte di una richiesta di euro 240.000. Si prevede che entro la fine dell'anno saranno accreditati alla corte d'appello di Firenze ulteriori fondi per circa euro 28.500.

Si prevede che entro la fine dell'anno saranno accreditati ulteriori fondi per circa 14.300 euro. Per le spese postali,

dalla legge finanziaria, verranno assegnati ulteriori accreditamenti. Per quanto riguarda le spese per l'acquisizione di riviste e pubblicazioni giuridiche, le risorse allo stato stanziate sono irrisorie rispetto alle richieste per soddisfare almeno in parte le esigenze degli uffici ma compatibilmente con lo stanziamento di cassa saranno disposti ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati. Analogo critico problema riguarda il parco auto e i fondi assegnati ai funzionari delegati, che sono competenti per territorio e operano in regime di discrezionalità.

al tribunale di Lucca sono state assegnate un'autovettura a noleggio e due autovetture ordinarie di proprietà. Alla procura della Repubblica di Lucca sono assegnate un'autovettura in noleggio e un'autovettura ordinaria di proprietà. In conclusione, si rappresenta che gli stanziamenti previsti per l'anno 2007 nel disegno di legge di bilancio preventivo non presentano significativi aumenti rispetto agli stanziamenti dell'anno 2006. Tuttavia, disegno di legge finanziaria predisposto per l'anno 2007, si delinea un'inversione

Invero, è stato previsto un fondo straordinario che in gran parte assorbe le decurtazioni *ex* legge di conversione del decreto Bersani per 200 milioni di euro, da destinare alle spese dell'organizzazione giudiziaria, della giustizia minorile e dell'amministrazione penitenziaria. In virtù della disponibilità di questo fondo, sarà possibile utilizzare una parte dello stesso per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le quali rientrano tra le spese relative all'organizzazione giudiziaria.

Tuttavia mi preoccupa la previsione che nel 2007 la situazione non sarà molto diversa. Mi preoccupa nel senso che è bene che lo stesso Parlamento sia stato puntualmente informato e possa insieme al Governo trovare una soluzione. la mia insoddisfazione, ovviamente soprattutto rispetto al lavoro che i suoi uffici hanno compiuto? Alla fine dell'interrogazione il senatore Caprili e io manifestavamo

una strada per sospendere il vecchio ordinamento giudiziario approvato nella precedente legislatura, e si è data dei tempi per realizzare una riforma, anche tenendo conto di tutto ciò che il Parlamento ha già costruito. Ecco quindi il punto. Noi usciamo da una fase importante, quella di una discussione dell'Assemblea del Senato, anche con convergenze su alcuni punti tra maggioranza e opposizione, sul tema di una giustizia più rapida e più giusta; avremmo voluto che il Governo, al di là dell'aspetto numerico, esprimesse

e ritengo opportuno che da parte dei presentatori di questa interrogazione si definisca una proposta organica tesa a risolvere tali problemi (che, al di là della carenza di risorse, in noi grande preoccupazione), affinché nella Provincia di Lucca, ma in generale in tutto il Paese, la giustizia sia sempre più rapida e più giusta e quindi una giustizia moderna.